i due incaricati di commemorare domani Garibaldi, perché, tra l'altro, sono due miei vecchi amici. Tuttavia, signor Presidente, mi chiedo come mai la commemorazione di Garibaldi nell'Aula del Senato avvenga soltanto ad opera di un membro del Governo e di un componente della maggioranza: Garibaldi, signor Presidente, è patrimonio storico di tutti noi. Le faccio presente questa mia osservazione perché eventualmente consideri l'opportunità che anche qualcuno dell'opposizione possa commemorarlo.

deliberato dalla Conferenza dei Capigruppo la settimana scorsa e comunicato all'Assemblea, prevede per la giornata di domani l'avvio della discussione del provvedimento sull'ordinamento giudiziario, esame si è concluso presso la Commissione giustizia pochi minuti fa. A margine del calendario vi era anche la scadenza per le ore 19 di oggi del termine per la presentazione degli emendamenti.

prevista per domani, sia stata invitata la famiglia Garibaldi, ricordando che l'ultimo degli eredi è il dottor Giuseppe Garibaldi, pronipote diretto del generale Giuseppe Garibaldi. Mi auguro che il Senato abbia invitato la famiglia Garibaldi e il pronipote che è vivente. **Sui

approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario fino al 14 luglio. La seduta pomeridiana di oggi - come già previsto dall'ordine del giorno - è dedicata alle repliche di relatore e Governo e alle votazioni degli emendamenti e degli articoli del disegno di legge in materia fiscale, con l'auspicio di concluderne l'esame. Ove ciò non fosse possibile, la trattazione riprenderà a conclusione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario. Resta confermato che la discussione generale della riforma dell'ordinamento giudiziario si svolgerà nel corso di questa settimana secondo le scansioni già previste dal calendario vigente. La discussione generale medesima si concluderà nella seduta antimeridiana di martedì 10 luglio. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 19 di domani. Le votazioni sul provvedimento avranno inizio dalla seduta pomeridiana di martedì 10 luglio e proseguiranno nelle giornate successive, al fine di pervenire alla votazione finale entro la giornata dì venerdì 13 o - se necessario - nella seduta antimeridiana di sabato 14. Il voto sulle dimissioni dei senatori Vernetti, Magnolfi e Selva avverrà all'inizio della seduta pomeridiana di domani, anziché a fine mattinata come precedentemente indicato. Rimane all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di giovedì 5 luglio il disegno di legge, fatto proprio dalla Lega, recante delega per la nomina elettiva dei giudici di pace, con l'avvertenza che, ove la trattazione del provvedimento dovesse concludersi prima delle ore 11,30, si passerà in ogni caso al seguito della discussione generale sull'ordinamento giudiziario anche prima di tale orario. Se l'*iter* dell'ordinamento giudiziario lo consentirà, alla fine della prossima settimana sarà avviata la discussione del decreto-legge in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia. Nel corso della Conferenza dei Capigruppo è emersa l'esigenza di comunicazioni del Governo sul rapimento del missionario italiano nelle Filippine, padre Giancarlo Bossi. La Presidenza si è già attivata per acquisire la disponibilità del Governo al fine di dedicare al più presto uno spazio a tale dibattito. Avverto, infine, il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 5 luglio, alle ore 12,15, per il sesto scrutinio relativo all'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi i deputati. La chiama dei senatori avrà inizio orientativamente attorno alle ore 14.

nelle Filippine dalla sua nativa Abbiategrasso, il «gigante buono» - come veniva e viene chiamato - vive ed opera nell'isola di Mindanao, l'unica zona non cattolica delle Filippine, «al servizio e per l'assistenza morale e fisica del prossimo più bisognoso», come ha scritto il presidente Cutrufo in una lettera indirizzata al ministro D'Alema. Il 10 giugno, al termine della celebrazione della Santa messa, un manipolo di dieci uomini lo ha caricato su un battello ed è svanito nel nulla, anche se è stato fatto sapere che è in buone condizioni fisiche. Sabato scorso, in un articolo di fondo del «Corriere della Sera», dal titolo «L'ostaggio dimenticato», si evidenziava la terribile percezione di ingiusta disparità nei confronti di altri casi di sequestri di nostri connazionali. È una terribile percezione che purtroppo sembra non infondata. Sono peraltro convinto che, data la delicatezza e la riservatezza che deve sempre esserci nella gestione dei rapimenti, la nostra diplomazia stia mettendo in atto quanto necessario con la consueta capacità: un impegno senza risparmio e senza riserve per salvare la vita di chi si trova nelle mani di fanatici senza scrupoli. Il Governo allora deve fugare questa terribile percezione e la deve fugare, come lei ha detto, signor Presidente, pur nell'ambito della necessaria riservatezza, di fronte al Parlamento. Il Governo in Parlamento deve correggere la terribile sensazione che il proprio impegno politico, anche ai livelli più elevati, per la liberazione di padre Giancarlo Bossi stia avvenendo con minore determinazione rispetto ad altri casi. Chiedo - e sono contento che lei abbia già dato questa assicurazione - che, senza che, senza polemica e senza strumentalizzazione alcuna, di fronte all'assoluta esigenza di salvare una vita umana e nel dovuto rispetto delle nobilissime parole

Signor Presidente, sarò brevissimo. Ho ascoltato gli interventi in discussione generale e mi riservo di dare risposte in occasione dell'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti. Sottolineo che si tratta di un provvedimento di particolare importanza, atteso dalle categorie e dai contribuenti.

ad alcune di esse ci sono addirittura documenti parlamentari che chiedono al Governo di procedere con strumenti d'urgenza, anche con decreti-legge.

Comunico che sono stati ritirati i seguenti emendamenti:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo con l'osservazione che, stante l'avvenuto rinvio del termine per la presentazione delle istanze di rimborso dell'IVA, appare necessario che il Governo fornisca gli adeguati elementi informativi sui relativi andamenti in materia di rimborso. In ordine agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100, 1.101, 1.102, 1.103,

Esprime poi parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.101, 2.102 e 2.103. Esprime, altresì, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla eliminazione del comma 2, sulla proposta 2.0.113. Il parere non è ostativo sulle restanti proposte emendative, fino all'emendamento 2.0.118 a partire dal quale l'espressione del parere è rinviata». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.118, 2.0.119,

Esprime inoltre parere di semplice contrarietà sulle proposte 6.0.100, 6.0.101 e 6.0.102. Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte emendative, ad eccezione che sugli ulteriori emendamenti per i quali l'espressione del parere è rinviata». rinviata». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.0.500, esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.0.1 (testo 2). Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte emendative, ad eccezione degli emendamenti

l'ordine del giorno G111 del senatore Eufemi, mentre esprimo parere contrario sulla premessa e sul primo periodo del dispositivo, parere favorevole al secondo periodo del dispositivo, che recita: «A dare completa attuazione del Protocollo sugli studi di settore e sviluppo economico, recuperando un più forte clima di fiducia con le categorie produttive».

come giustamente ha esposto il relatore, il contenuto dell'ordine del giorno a mia firma è stato trascritto quasi integralmente nella mozione già approvata dalla maggioranza. Sono anche in discussione degli emendamenti per renderne ancora più stringente il contenuto. Ciò considerato, accolgo l'invito al ritiro.

avevamo presentato questo ordine del giorno ben prima dell'esame in Aula della vicenda degli studi di settore e avevamo visto giusto. Ora, come si fa a dire no a tutta la premessa quando essa è la ricostruzione degli avvenimenti? Noi poniamo il problema della piccola e media impresa, che viene particolarmente colpita rispetto a un'elevata pressione fiscale. Con gli indicatori di normalità economica è stato costruito un mondo è stato costruito un mondo virtuale non corrispondente alla reale normalità economica. Come si fa a negare che è stato sperimentato, nel caso del catasto rurale, un aggiornamento errato della banca dati del catasto terreni, che ha comportato anomalie ed errori tali da dover essere corretti in questo provvedimento? Infatti, sono state effettuate riclassificazioni in qualità colturali superiori, con conseguente lievitazione delle rendite. Presidente, non mi sorprendo che la maggioranza presenti dieci ordini del giorno, che contengono altrettante indicazioni

primo riguarda in particolare il significato degli indicatori. Così come recita la mozione del Senato, gli indicatori hanno un carattere che non inverte l'onere della prova, ma lascia all'Amministrazione

ribadiscono l'entrata in vigore degli studi di settore dal 1° gennaio 2007, allora l'ordine del giorno è pleonastico e non si capisce la ragione per la quale non debba essere recepito. Altra questione: nella premessa viene ribadita l'esigenza di un forte contrasto all'evasione fiscale, alla concorrenza sleale, alla contraffazione, al lavoro irregolare e a quant'altro. Aggiungo ancora che la questione della sperimentalità è di tutta evidenza e ribadisco ciò che la stessa senatrice Thaler Ausserhofer aveva sostenuto in Commissione ovvero che gli studi di settore non hanno tenuto conto degli elementi contingenti relativi all'ubicazione

a un disegno di legge riguardante temi importanti, soprattutto - come ho detto in discussione generale e ribadisco - quello degli ammortamenti, come correzione di errori gravissimi che avevano generato anche nel settore immobiliare un danno molto rilevante ai tempi della stesura stesura della norma originaria. Ma vedo che questa schizofrenia nella gestione della politica fiscale evidentemente continua, perché non ci si mette nelle condizioni di fare delle valutazioni appropriate

cui destinazione a breve vedremo in un decreto-legge del Governo, secondo quanto scritto all'interno del Documento di programmazione economico-finanziaria.

luogo bocciando gli emendamenti che già in Commissione noi come Lega Nord, ma anche altri colleghi, avevamo proposto, che andavano nella direzione di accogliere le giuste rimostranze fatte dalle associazioni degli imprenditori al Presidente del Consiglio e al ministro Bersani nelle assemblee che conosciamo.

(cosa tutta da verificare, perché mi risulta che non tutte le associazioni abbiano poi dato il via libera, l'ok a questo accordo con il vice ministro Visco, quindi, a maggior ragione, la sospensione che avevo proposto era fondata in quanto il lavoro per risolvere questo problema è *in itinere*), andremo ad approvare degli emendamenti limitativi - probabilmente approvati solo per spirito di disciplina di maggioranza, di corpo - senza discutere di un problema così importante e fondamentale.

Per questo motivo, quindi, ho fatto miei, come Gruppo, gli emendamenti della senatrice Thaler Ausserhofer, proprio allo scopo di votarli e di far emergere a questo punto non solo la schizofrenia, ma anche l'incoerenza di chi, all'interno della maggioranza, propone delle soluzioni concrete che vanno nella direzione di dare risposte all'impresa italiana, che dopo vede ritirati questi emendamenti ai quali seguono seguono delle ulteriori proposte, probabilmente - io spero che non sia così - raffazzonate, che poi non saranno quelle che corrisponderanno al definitivo e concluso accordo fra il Governo e le parti sociali.

del peggio del peggio è meglio solamente il peggio), ma sulle quali effettivamente una discussione, una seria proposta, un confronto con le parti sociali

non esagerate, serie e concrete su alcuni temi specifici e vedremo di inserirle; perché un grande richiamo da parte del mondo dell'imprenditoria a queste risposte era stato era stato fatto, c'era stato comunicato, c'era stato illustrato in diversi modi; quindi sto parlando anche di altre questioni non solamente quelle che riguardano gli studi di settore. Per questo abbiamo presentato alcuni emendamenti

«In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione

finanziaria. Riguarda la posizione patrimoniale di decine di migliaia di famiglie e di piccoli imprenditori i quali, già sottoposti ad una vessata tassazione

Pertanto, con l'emendamento 1.1 si vogliono escludere effetti indiretti di retroattività determinati dalla formulazione finale della disposizione indicata Per effetto di quella norma, infatti, con riferimento ai fabbricati strumentali acquistati prima del periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006, il fondo di ammortamento dedotto in precedenza sarà riferito proporzionalmente al costo del terreno e a quello della costruzione che insiste sullo stesso mentre in precedenza era previsto che il fondo fosse imputato prioritariamente al costo di fabbricato. In sostanza, il fondo di ammortamento viene riferito *pro quota*, distintamente, sul terreno e sul fabbricato. Questa norma ha evidentemente riflessi positivi per le imprese, anche in riferimento agli immobili acquisiti in *leasing* sulla base di contratti stipulati antecedentemente al 2006. Poiché la norma entrerà in vigore quando la maggior parte dei bilanci di impresa relativi al 2006 saranno già definitivi, e quindi non potranno più essere modificati, vuole introdurre un regime transitorio che consenta di recuperare fiscalmente gli ammortamenti non dedotti nell'esercizio nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero nell'esercizio stesso e in quelli successivi. La norma che si propone non produce effetti di minore gettito rispetto a quelli originariamente stimati in sede di relazione tecnica poiché la quantificazione, basata peraltro su dati macro di bilancio non relativi al singolo fabbricato e al suo stadio di ammortamento, in conformità con l'intento perseguito non teneva conto dell'effetto penalizzante che ho appena descritto. Pertanto, alla norma proposta non è ascrivibile alcuna perdita di gettito rispetto alla stima contenuta nella relazione tecnica e quindi noi non ci riconosciamo nel parere che è stato espresso dalla Commissione bilancio.

perché naturalmente ha portato all'emersione del lavoro nero, del sommerso, nell'ambito delle costruzioni. Noi riteniamo che la proroga del 36 per cento debba essere allargata anche agli immobili abitativi ristrutturati dalle imprese e non dal singolo. Infatti molte volte il singolo rinuncia per la complessità delle procedure, per la complessità degli oneri burocratici e preferisce non utilizzare questa procedura piuttosto che imbarcarsi in qualcosa di complesso. Le Le imprese di costruzioni, invece, molte volte agiscono sulla ristrutturazione complessiva e possono poi presentare al singolo utente un'operazione già definita.

proponiamo di rinviare la definitiva applicazione delle norme sull'accertamento, in base al valore normale, alla data di entrata in vigore del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che definirà i criteri oggettivi, attribuire efficacia all'accertamento presuntivo, in ogni caso con riferimento ai trasferimenti immobiliari effettuati in data successiva al 4 luglio del 2006.

in via definitiva, che il regime agevolativo si intende applicabile ai trasferimenti diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, purché sia presente una quota di edilizia convenzionata, realizzata in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione di prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Abbiamo visto la crisi che si è determinata nei programmi di edilizia sociale e soprattutto in quella residenziale: vi è necessità di intervenire, di determinare le condizioni affinché i giovani, le giovani coppie possano acquisire degli alloggi perché oggi esiste una crisi dell'alloggio che non può essere sopperita soltanto con i prezzi di mercato e richiede, invece, anche un intervento dell'edilizia convenzionata. Per queste ragioni riteniamo che si debba insistere per l'emendamento 1.0.3.

una questione che abbiamo già affrontato in sede di Commissione, anticipata al relatore,

delle colture agricole - laddove gli ingegneri sono incorsi in un errore colossale perché non sono stati affiancati dagli agronomi e quindi hanno confuso il pomodoro industriale con il pomodoro da coltura ortiva - noi abbiamo sollevato un'altra questione che meriterebbe attenzione che è quella degli accessi nei fondi rustici, soprattutto nelle aree di montagna e nelle aree interne.

il conduttore agricolo ne paghi soltanto uno, anche a fronte delle esigenze di sicurezza che vengono portate avanti favorendo questa soluzione. Presidente, naturalmente avrei ancora molte altre cose da dire, mi sono limitato a quattro o cinque punti essenziali, sui quali richiamo l'attenzione di quest'Aula affinché questo provvedimento non sia soltanto una correzione marginale, ma qualcosa di più significativo.

i quali hanno fatto propri a nome dei loro Gruppi, e mi accingo a fare lo stesso per il Gruppo di Forza Italia, gli emendamenti ritirati dalla senatrice Thaler di emendamenti che, con intensità diversa, perseguono tuttavia tutti obiettivi di contenimento dell'azione condotta dal vice ministro Visco in spregio agli elementari diritti del contribuente. Essi, per esempio, si rivolgono alla non retroattività di molte misure; in modo particolare, per quanto riguarda gli studi di settore, tali emendamenti ripropongono il tema della loro non retroattività e quello della non inversione dell'onere della prova nel caso di accertamenti connessi agli scostamenti che nelle dichiarazioni dei redditi si dovessero registrare rispetto alle soglie degli studi di settore, così come modificati dagli indicatori di normalità. Invero, nel corso di questi giorni il vice Ministro ha aggiunto confusione a confusione, aggravando l'incertezza dei contribuenti e delle attività professionali che li assistono. In un primo momento, il vice ministro Visco ha accettato la natura sperimentale di questi nuovi indicatori che, tuttavia, nulla toglie al loro effetto repressivo; successivamente, l'Amministrazione finanziaria e il Vice ministro stesso hanno parlato di non automaticità dell'accertamento, così come si affermava nella mozione approvata dalla maggioranza. Ma anche in questo caso nessuna novità, in realtà, veniva introdotta con riferimento agli studi di settore modificati dagli indicatori di normalità.

si determina l'accertamento con inversione dell'onere della prova; oggi un'ultima dichiarazione unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze afferma che vi sarebbe un'intesa con alcune organizzazioni circa la non inversione dell'onere della prova per tutti gli accertamenti che diventerebbero pertanto accertamenti semplici e non da studio di settore.

tale è la natura sostanziale di queste norme retroattive che il Governo, in sede di legge finanziaria, ha attribuito ad esse uno specifico effetto finanziario, nella misura di 2,6 miliardi di euro. Pertanto, nel momento in cui venisse meno l'effetto della deterrenza, determinato dall'inversione dell'onere della prova, connesso cioè all'accertamento da studio di settore, verrebbe ragionevolmente meno anche, in tutto o in parte, l'effetto finanziario specifico

Per queste ragioni noi vorremmo, in realtà, che il Senato cogliesse l'ultima opportunità che ha di fermare quest'atto di inciviltà giuridica, consistente nell'introduzione, con effetto retroattivo, di norme sostanziali che auspicano

consona. Questa mattina, prima dell'inizio della seduta, la senatrice Thaler ed altri colleghi hanno ritirato i loro emendamenti. Iniziata poi la seduta, si è preceduto come tutti sappiamo e, ad un certo punto, i colleghi della Lega hanno chiesto di far propri gli emendamenti presentati dalla senatrice Thaler e ritirati prima dell'inizio dei lavori

l'articolo 100 del nostro Regolamento, al comma 13, prevede, in maniera esplicita e netta: «Gli emendamenti sono di regola stampati e distribuiti in principio di seduta». Quindi, l'inizio della seduta è il momento nel quale c'è la notorietà degli emendamenti. Si considerano pertanto emendamenti quelli presentati prima dell'inizio della seduta: perciò, se prima dell'inizio della seduta un emendamento è stato ritirato e non c'è più, non può essere

prima dell'inizio delle votazioni e prima della seduta, correttamente, un emendamento può essere ritirato. Presidente, mi pare logico, oltre che rispettoso del Regolamento, che se un emendamento viene ritirato prima dell'inizio della seduta non possa essere esaminato in Assemblea. se il titolare dell'emendamento ha la volontà di non presentare all'Assemblea il suo emendamento, tant'è che lo ritira prima dell'inizio della seduta, il Presidente dell'Assemblea e l'Assemblea stessa non possono esaminarlo dal momento che non esiste più perché il presentatore lo ha ritirato

Se fosse vero il contrario, nascerebbe un problema di una certa gravità: quand'è che cessa il diritto del senatore di

che la Presidenza debba tener conto anche di queste osservazioni e, se del caso, chiedere alla stessa Assemblea un parere. Infatti, trattandosi di una questione di enorme rilevanza, che modifica la vita e le procedure parlamentari lasciando nel limbo la possibilità di ritirare o meno gli emendamenti in quanto non ci sarebbe una scadenza fissa,

punto, il diritto del senatore prevale su tutto, perché è in quel momento che il senatore viene a sapere che l'emendamento è stato ritirato. Se non accettiamo questa impostazione,

Allora, innanzi tutto la Presidenza deve essere attenta al rispetto di un diritto sostanziale del singolo senatore; semmai lei mi potrà obiettare: organizziamo i lavori del Senato per cui un minuto prima della apertura della seduta si ristampi

Questa è la ragione di fondo che mi fa sostenere, in relazione alla nostra prassi, che non posso togliere il diritto al senatore Franco Paolo di farli propri perché è venuto a conoscenza di questo. Farò studiare agli Uffici la possibilità di un aggiornamento dello stampato anche dieci minuti prima

facoltà. CALDEROLI *(LNP)*. Io credo che il senatore Boccia avrebbe perfettamente ragione fin tanto che non si arriva al momento della prima stampa degli emendamenti. Nel momento in cui l'atto è diventato pubblico, deve essere comunicato all'Assemblea se è cambiato qualcosa.

rimanesse agli atti dell'Assemblea in maniera chiara: gli emendamenti quindi possono essere ritirati prima che sia stampato il fascicolo. Questa è la decisione della Presidenza?

Signor Presidente, al di là della questione puramente tecnica, l'intervento del senatore Boccia dimostra, ove ve ne fosse bisogno, l'imbarazzo non solamente del Governo, ma anche della maggioranza rispetto a questo problema. Quindi, molto opportunamente, i colleghi Franco ed Eufemi hanno ritenuto di non far disperdere nel vuoto l'iniziativa meritoria fino ad un certo punto della collega Thaler che va in direzione di un'equità fiscale che intendiamo ribadire in questa sede e rivendicare. Rispetto agli studi di settore si è consumato un autentico mostro giuridico, attraverso l'introduzione del principio della retroattività delle norme fiscali e tributarie, che credo rappresenti il livello più basso di inciviltà giuridica e politica in termini economici perché si riversa sostanzialmente su alcune categorie di contribuenti che oggi sono particolarmente vessati dalle imposizioni fiscali. È questo il motivo per cui anche il Gruppo AN ritiene opportuno che questo disegno di legge, giustamente definito urgente, abbia bisogno però di una valutazione complessiva perché da questo provvedimento vorremmo evincere quale è la linea di politica fiscale e tributaria di questo Governo; una linea fino a questo momento assolutamente non chiara, sicuramente molto ambigua, certamente vessatoria, così come è dimostrato anche dagli ordini del giorno presentati dai colleghi della maggioranza, che noi abbiamo la volontà di fare emergere all'interno dell'Assemblea. Ecco perché, insieme ai colleghi Franco ed Eufemi,

la necessità di introdurre un'imposta sostitutiva del 20 per cento sulle plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di beni immobili, acquistati o costruiti da meno di cinque anni, e di terreni agricoli suscettibili di utilizzazione edificatoria.

tenendo conto che il Governo ha accolto un ordine del giorno che pone la necessità di confermare

1.0.5 perché è stato già approvato in Commissione e ora in Aula un ordine del giorno che fa propria l'indicazione da lui richiesta per via emendativa.

riconferma in questa occasione le posizioni già espresse in occasione della discussione e della votazione del decreto-legge fiscale

con una politica di contrasto all'evasione fiscale. Infine, esprimo parere contrario agli emendamenti 1.0.101 e 1.0.102

con i quali risolviamo problemi importantissimi per i contribuenti, per i piccoli imprenditori, ho ritirato tutti gli altri emendamenti. Dichiaro pertanto che mi asterrò dalla votazione su tutti gli emendamenti da me ritirati

FI)*. Ma se le previsioni tecniche erano sbagliate e abbiamo trovato un tesoretto, anzi un dividendo Tremonti, come lo abbiamo

che, quando modificammo il Regolamento, per fare in modo che non questo o quell'emendamento, ma tutti gli emendamenti che ricevono parere contrario della 5a Commissione in base all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,

tutelare l'applicazione corretta dell'articolo 81 della Costituzione, anche dopo che il Parlamento abbia deliberato su una legge. Per tale motivo,

nel merito. Naturalmente, il Parlamento può votare un emendamento scoperto, ma deve sapere che lo sta facendo e che sta così determinando una situazione di particolarissima gravità. Per questo motivo, abbiamo modificato il Regolamento in tal senso. Io quindi insisto: secondo me, non bisogna accettare dichiarazioni di voto su emendamenti improcedibili,

Presidente, l'approvazione dell'emendamento 1.100 crea problemi ad un provvedimento che era tutto a vantaggio dei contribuenti e delle piccole imprese;

Grazie, Signor Presidente, vorrei ricordare che questo provvedimento contiene disposizioni - e gli emendamenti ad esso relativi ne aggiungono altre - che hanno a riferimento le dichiarazioni dei redditi per le quali sono prossime le scadenze. Chiedo, pertanto, di procedere ad oltranza fino all'approvazione definitiva del provvedimento.

l'approvazione dell'emendamento che sostituisce integralmente l'articolo 1 pone la necessità di una valutazione da parte della Commissione.

disegno di legge, non costituisce ostacolo a che si possa proseguire nella votazione e nella discussione degli emendamenti aggiuntivi. Chiedo solamente che ci sia - come eravamo rimasti d'intesa - allorché arriveremo all'esame dell'articolo 2, la possibilità per la Commissione bilancio di esprimere il parere su sette emendamenti sui quali si era riservata di svolgere le sue valutazioni.

il senatore che vota anche per un collega assente normalmente lo fa all'ultimo secondo, proprio nel momento in cui lei dichiara chiusa la votazione; è quello il momento in cui il senatore assente risulta improvvisamente tra

ci sia effettivamente il senatore, perché in questo caso ciò è avvenuto e noi non siamo in condizioni di impedirlo. *(Commenti del un po' anomalo che si prenda la parola non al momento in cui si verifica il fatto, o comunque si ritiene che si verifichi il fatto,

è il comportamento di alcuni componenti della maggioranza, se non - considerato che gli altri non hanno parlato - della maggioranza stessa. Vorrei sapere come ha speso il suo tempo la maggioranza in questa mezz'ora:

che o il vice ministro Visco se ne va, e questa volta per ragioni di carattere politico e non per altre, oppure è la vostra maggioranza che non è più tanto coesa da riuscire a sostenere la politica del vice ministro Visco. Quindi, non nascondetevi dietro ai voti espressi e che per caso sono stati tolti.

Presidente, credo abbia ragione il collega Paolo Franco nel momento in cui rileva che, al di là delle osservazioni capziose relative al funzionamento del sistema elettronico, è emersa manifestamente una questione fiscale che, in certa misura, tocca anche i settori della maggioranza. Quell'emendamento, come molti altri a prima firma della senatrice Thaler, che hanno contenuti analoghi a quelli presentati dall'opposizione, era rivolto ad eliminare aspetti odiosi, relativi soprattutto alla retroattività di molte disposizioni fiscali contenute in vari provvedimenti, tra i quali, come in questo caso, il famigerato decreto Visco-Bersani. Credo soprattutto che salga dal Paese una forte pressione di cui anche alcuni esponenti della maggioranza si fanno portavoce, fermandosi tuttavia alla soglia del voto, com'è accaduto poco fa

tutti coloro i quali saranno interessati ai trasferimenti di questi immobili, soprattutto dei suoli edificatori, applicando su questo trasferimento un'aliquota giusta del 20 per cento, dichiareranno tutti il prezzo reale sulle vendite degli immobili.

e tutti i colleghi anche dell'opposizione a votare a favore di questo emendamento perché introduce un'aliquota giusta su un

Presidente, quando un'Aula del Parlamento approva un emendamento, ancorché non condiviso dalla maggioranza e con i problemi di registrazione del voto che sono emersi, la cosa più elementare è prendere atto che c'è stato un risultato non desiderato, non previsto, né desiderabile;

prevalentemente - per non dire esclusivamente - gli interessi politici di parte, la possiamo raccontare come

il *deficit* di previsione di entrata o il *deficit* di spesa pubblica di un "x" o di un "x" più un possiamo utilizzare anche questo argomento per dire che i conti fatti da questo Governo sono sbagliati e le previsioni saranno disastrose. Tuttavia, una cosa è certa, vale a dire che che era stato votato in Commissione, prevedeva la possibilità per gli imprenditori e i proprietari di aree agricole e fabbricati di poter calcolare l'ammortamento su questi beni, mobili e immobili, con un meccanismo capace di costituire, da una parte, una risposta positiva a una sollecitazione in questi termini omogenea da parte dell'Unione Europea, che indica un criterio di ammortamento;

rappresentava un beneficio per il proprietario, che era assolutamente previsto, prevedibile e quantificabile. Con l'approvazione dell'emendamento sostitutivo abbiamo determinato una condizione per la quale ciò che

se c'è qualcosa che non va sono pronto a discuterne!

il meccanismo del lotto convenzionato tra lo Stato e le società, si determinano problemi a catena di cui le società convenzionate non si fanno carico e non intendono ovviamente farsi carico. Credo

degli immobili, di cui all'articolo precedente, con un ulteriore incremento del prelievo sulle vincite al lotto dal 6 al 10 per cento, cioè di altri quattro punti.

negoziare politicamente un determinato risultato, queste previsioni, che pur non sono ragionevoli né razionali, possono trovare una giustificazione politica molto forte e consolidata. Tuttavia, nel momento in cui

diversificate, con l'intenzione e l'obiettivo di arrivare ad una revisione della norme adottate in precedenza, che avevano suscitato una reazione legittima da parte delle categorie e che, a fronte delle intese raggiunte tra le associazioni ed il Governo, possono trovare negli emendamenti sui quali la 5a Commissione ed il Governo si pronunceranno appena possibile

che con l'emendamento votato poc'anzi e approvato dall'opposizione, diventata maggioranza, abbiamo incrementato l'imposta sui giochi del lotto. Si è incrementata la ritenuta delle vincite: una cosa molto diversa, come tutti sanno. sanno. Bisogna evitare di far credere che con l'emendamento appena approvato si sia, per così dire, danneggiata l'idea dello Stato biscazziere. Non so se questa maggioranza si sia ormai decisamente orientata all'idea dello Stato biscazziere per reperire fondi. Certo, di cose illegittime ne fa tante, ma lo Stato biscazziere da questo punto di vista non c'entra.

a "Porta a Porta", a "Ballarò", a "Matrix" l'onorevole Rutelli affermare più volte - mai ascoltato dalla sua maggioranza e non so se lo sarà adesso,

sul reddito degli immobili in modo da recuperare una fascia di evasione notevole senza il rischio di pagare di più dal punto di vista dell'IRPEF: esattamente l'emendamento Girfatti. Delle due l'una: o le affermazioni di Rutelli lasciano il tempo che trovano, sono parole dette in libertà e la parte della maggioranza che dice di riconoscersi in lui non le vuole far proprie perché preferisce l'ipotesi dello Stato biscazziere - prenderemo atto,

Stiamo lavorando per evitare che i cosiddetti tesoretti si formino da una eccessiva tassazione imposta agli italiani. Volete continuare a far finta di parlare di tesoretti o continuare nella linea

la teoria secondo la quale Visco rappresenta l'intera maggioranza o prende atto che Visco rappresenta se stesso, o poco più di se stesso, e si libera di questo peso iniziando una politica fiscale diversa? Questo è il senso dell'emendamento Girfatti.

Signor Presidente, per la verità non ho la stessa sicurezzadel senatore D'Onofrio sul merito di questo emendamento, anzi, ho un'opinione radicalmente opposta. Ne avevamo discusso anche in Commissione in Commissione e avevamo manifestato le perplessità che cerco ora di rappresentare ed esplicitare. In realtà, l'emendamento

perché costituisce una occasione ed una opportunità messa a disposizione sopratutto di chi può essere nella condizione, grazie a quel meccanismo fiscale poi introdotto, di ricevere un particolare beneficio ed una particolare remunerazione dall'investimento che va a realizzare. Se qualcuno avesse un po' di esperienza di ciò che succede nei Comuni, nei territori ed avesse un po' di esperienza di Governo delle problematiche urbanistiche, sarebbe consapevole o condividerebbe con me il fatto che questa norma potrebbe avere degli usi, delle applicazioni ed implicazioni del tutto distorsive dello sviluppo urbanistico di un territorio, di una comunità e premiare e privilegiare soprattutto coloro che rientrano nelle caratteristiche dei grandi operatori immobiliari e delle speculazioni dal punto di vista della crescita e delle modifiche di interventi urbanistici sui territori, nelle comunità e quant'altro. Da questo punto di vista, il riferimento ad un principio di armonizzazione al 20 per cento della transazione sugli immobili, che consideri anche la remunerazione degli affitti e così via, è tutt'altra cosa, nel senso che quello è un un criterio che auspichiamo di vedere gradualmente tradotto e reso come norma a vantaggio del contribuente per una misura di equità fiscale e sociale e anche per un incentivo alla trasparenza e all'emersione. Tuttavia, la norma, così come si presenta, è costruita in maniera da rappresentare un regalo - permettetemi questa espressione - fatto a possibili grandi interventi ed interessi di speculazione immobiliare e terriera e certamente non va nella direzione né della lotta all'elusione e all'evasione, né del privilegio e nell'attenzione alla generalità dei contribuenti; certamente è una norma che va esattamente nel senso opposto allo spirito e l'intenzione di questo provvedimento, proposto all'attenzione ed al lavoro dell'Assemblea

da respingere, perché, oltre che avere riflessi onerosi già richiamati nell'intervento del senatore Bonadonna, ha ovviamente anche quegli aspetti di merito, su cui ho cercato di soffermare la mia attenzione, particolarmente importanti e delicati, perché possono costituire un *vulnus* al Governo del territorio, alla correttezza dello sviluppo delle nostre città ed ai piani ed ai programmi di edificazione, che insistono sui diversi contesti urbani territoriali.

della detrazione IRPEF del 36 per cento in relazione alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare. la disposizione che prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili abitativi. Questa aliquota ridotta è in linea anche con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea. signor Presidente, che questo emendamento possa essere approvato, perché la combinazione di questi elementi che ho richiamato determina effetti positivi sia in termini di recupero dell'evasione, che in termini di incremento dell'occupazione e degli investimenti in tali settori...

Queste sono le ragioni per le quali prevediamo di estendere la proroga del 36 per cento anche all'acquisto degli immobili abitativi ristrutturati dalle imprese. Si possono massimizzare gli effetti positivi con misure che hanno dimostrato ampiamente una loro validità sin dalla loro istituzione. Voglio ricordare

perché ha voluto ostinatamente rifiutare qualsiasi emendamento, qualsiasi azione positiva proveniente dall'opposizione

se quanto contenuto nel comunicato del Consiglio dei ministri dei primi di giugno sia stato tradotto in un atto

Per queste ragioni, Presidente, insisto per la votazione

ascoltare me? Vorrei interloquire con il collega Eufemi, anche perché questo argomento, oggetto del suo emendamento, è stato già discusso in Commissione

particolare. Nel merito, abbiamo ragionato sull'opportunità che un argomento di questa natura, invece di essere collocato forzosamente nel nel provvedimento al nostro esame, trovasse una collocazione più adeguata, magari nella prossima legge finanziaria, anche perché ad essa, si sta discutendo di misure legate al trattamento fiscale della casa, quindi della politica della casa.

So per certo che la sensibilità del collega Eufemi coincide sostanzialmente con la mia. Capisco che ci sono ragioni di battaglia politica che determinano un

una misura sulla politica abitativa, sugli sgravi per l'edilizia residenziale pubblica, sulle agevolazioni per coloro che mettono la casa in affitto e per gli inquilini che pagano che pagano affitti assolutamente esosi e quindi potremmo, da parte di quest'Aula, dare una risposta positiva a una parte della popolazione che aspetta dei benefici. In questo modo, noi non diamo risposta alcuna a questa area, socialmente rilevante, che vive il problema dell'emergenza abitativa. Riteniamo, invece, di metterci l'anima in pace e di salvare la nostra coscienza perché abbiamo realizzato un'operazione di trasferimento di alcune quote di agevolazioni fiscali

registrato in Commissione, di ritirare questo emendamento e di discuterne assieme in una sede nella quale questa materia trovi un terreno propizio di collocazione.

e buoni interventi dei colleghi ostruzionistici della maggioranza. Signor Presidente, non so se sarò capace di farla sognare, ma credo proprio di no. Non ho questa ambizione, e neanche quella di interessare l'intero uditorio con le poche considerazioni di merito che cercherò di svolgere.

di un ordine del giorno che abbiamo approvato e che il Governo ha accolto, che va nella direzione di recepire il senso dell'emendamento che è stato qui proposto alla valutazione dell'Assemblea. Tuttavia, è di tutta evidenza che un provvedimento di questa complessità (che è, come profilo, tutto orientato verso esigenze di miglioramento della condizione di trattamento del contribuente) deve comunque misurarsi con problemi di compatibilità finanziaria e di equilibrio del quadro finanziario.

va nella direzione di favorire interventi di riqualificazione edilizia, di ristrutturazione e di recupero di edifici storici, di premiare anche il conflitto di interessi, quello, però, ristretto e limitato ad ambiti precisi, tra contribuente e fornitore. L'estensione di questa norma, *sic et simpliciter*, alla generalità delle situazioni che che comprendono anche interventi di imprese su interi edifici e palazzi mi pare che, pur essendo stata sperimentata con qualche risultato positivo in passato, un problema di compatibilità di carattere finanziario e di necessità di sostegni ed integrazioni di fonti di finanziamento che non è stato possibile risolvere nel momento della discussione e dell'approvazione di questo provvedimento. Si è, quindi,

valide e disponibili per interventi di sostegno ulteriore all'economia e allo sviluppo, possa essere eventualmente utilizzata e destinata.

poter far fronte alle necessità finanziarie che immediatamente porrebbero un vincolo di difficoltà e renderebbero inagibile e impraticabile l'equilibrio finanziario dell'intero provvedimento. In realtà, quindi, tale emendamento rivela una motivazione e un profilo di

sembra esprimere un'intenzione dichiarata di farsi carico di esigenze dei contribuenti,

venire incontro a esigenze di miglioramento del rapporto tra fisco, amministrazione tributaria, Governo e contribuenti, in questo caso coloro interessati nello specifico dal provvedimento in questione.

intendete ancora votare o continuate a fare ostruzionismo contro il vostro Governo per evitare che quest'Aula voti? Soltanto questo volevamo sapere, dal momento che è in corso

abbia esigenze di accelerazione per la brevità dei tempi entro cui va approvato. Ci chiediamo questo, senza alcuno spirito polemico, ma allo stesso tempo chiediamo chiarezza. Noi siamo pronti a votare; vorremmo adempiere al nostro ruolo ruolo e alle nostre funzioni, perché, poi, quando si sostiene che in Senato non si vota e non si lavora più, non ci si venga a dire che è l'opposizione che paralizza questo Parlamento.

di non preoccuparsi: se anche il ministro Di Pietro ha reso certe dichiarazioni, stia tranquillo che voterà sicuramente il provvedimento, perché sarà allineato e coperto. Sono i classici *ballon

Appurato lo stato dell'arte (mi rivolgo all'opposizione e alla maggioranza, perché in questo momento credo sia difficile comprendere come potranno successivamente

arrivassimo anche al punto di quegli emendamenti, dovremmo comunque sospendere i lavori, con la differenza che la Commissione bilancio non si sarebbe riunita e i pareri non li avremmo a disposizione neanche per domani. È possibile utilizzare un po' di buon senso?